sulla eventuale collocazione della nuova struttura ed autorità all'interno della Presidenza del Consiglio. Ho chiesto stamattina un rinvio alla seduta pomeridiana perché il Governo si è fatto carico di alcune osservazioni formulate dal senatore Li Gotti ed in parte dal senatore Casson, anche se non è intervenuto. In particolare, con la proposta di emendamento 3.100 il Governo ha inteso soltanto adeguare alle Convenzioni internazionali la disciplina in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Quindi, tale proposta non riguarda l'eliminazione della concussione per fatti che riguardano l'Italia.

la finalità della Convenzione, quella cioè di evitare che il privato che corrompe pubblici ufficiali stranieri o appartenenti ad organizzazioni internazionali possa invocare l'induzione esercitata da pubblico ufficiale come discriminante e non essere processato. Negli altri Paesi europei questa ipotesi non è accettata ed è per questo che l'emendamento 3.100 (testo 2), di cui chiedo la votazione è

che peraltro in questo momento non è in Aula: quindi mi rincresce di non poter interloquire direttamente con lei, come avrei voluto. Ho ascoltato le ragioni che la medesima ha posto a fondamento di tale ordine del giorno, però mi permetto di annunciare su di esso un voto motivatamente contrario, innanzi tutto per una ragione di coerenza, che in qualche modo mi è caro rivendicare.

si realizzò una specie di consenso tra l'allora maggioranza di centrodestra e l'opposizione di centrosinistra sull'istituzione di questo benedetto Alto Commissariato, a riprova del fatto che sulle cose sbagliate è frequente ed agevole che si verifichi il consenso tra gli opposti schieramenti.

con personale, dipendenze e strutturazione quanto più possibile articolata e finanziata, che avesse la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della corruttela nella pubblica amministrazione.

il primo dei doveri di chiunque sia preposto ad una certa branca della pubblica amministrazione è non solo di dare contezza della propria assoluta trasparenza,

Questo è il difetto, o uno dei difetti dell'Italia istituzionale e politica contemporanea. Quando non riusciamo ad affrontare un fenomeno deteriore della nostra società e a risolverlo con la prevenzione o con la repressione adeguata, inventiamo un organismo, a cui diamo l'orpello della suprema indipendenza e neutralità e quant'altre parole di cui ci innamoriamo, che a sua volta diventa quasi sempre una nicchia di inefficienza, di spesa, di sovrapposizione e di burocrazia: è un serpente che gode nel mordersi la coda.

che dovrebbero legittimarne la reistituzione. Mi permetto di essere nettamente meno benevolo di lui, meno ottimista sulle prospettive della reistituzione e di affermare che questa non è la strada giusta.

Personalmente, sono molto "legnoso" da questo punto di vista e mi piacerebbe che maggioranza e opposizione di qualsiasi timbro avessero e manifestassero con i fatti una volontà politica per cui chi sgarra in questo senso è fuori per sempre e irrevocabilmente da qualsiasi *munus* *publicum* e da qualunque incarico della pubblica amministrazione, a qualsiasi livello, e che anzi questo costituisca per lui anche un elemento negativo per ogni altro tipo di prospettiva. La pubblica amministrazione deve essere gestita e rappresentata con mani illibate. Non è un problema di moralismo, è un problema di moralità diffusa e il senso dello Stato si manifesta prima di tutto su questo terreno. Molte colpe sono state accumulate da questo punto di vista. Mi permetto di dire, senza minima ombra di qualunquismo (che, lo sapete, mi è lontano un bel po'), che se negli ultimi negli ultimi 20-30 anni avessimo dato segnali precisi da questo punto di vista, oggi il tanto esecrato fenomeno di distanziamento dell'opinione pubblica rispetto alle istituzioni e la caduta della credibilità di queste ultime sarebbe

pertanto voterò contro per queste precise motivazioni, non di tenerezza verso la corruttela, ma anzi invocando assoluta inflessibilità da questo punto di vista. Mi permetterà anche di dire che, nel momento in cui parliamo di diminuzione degli organici di ogni organo ad ogni livello, di diminuzione del numero dei parlamentari, spesso credendoci e spesso facendone uno strumento, e

se i dipendenti siano 50 o 48 o 56, se dopo si lamenta l'insufficienza dell'organico (perché sempre si lamenta l'insufficienza dell'organico rispetto alle missioni che vengono conferite),

chiedo che si faccia occasione preziosa di questo tipo di confronti perché si manifesti con i fatti e non a parole la a parole la volontà di stroncare ogni possibile spazio del malcostume nella pubblica amministrazione. Per il resto, mi pare che il Governo, con l'intervento del Sottosegretario, abbia chiarito le preoccupazioni riguardo ai titoli di reato che venivano coinvolti da questa normativa. L'emendamento presentato dal Governo si allinea all'esigenza europea di intervenire sulle fattispecie delittuose e non vi è la benché minima intenzione di risparmiare la concussione

risponde ad un'esigenza precisa di dare attuazione all'articolo 6 della Convenzione che stiamo per ratificare, in quanto è previsto esplicitamente che ciascun Governo che ratifichi la Convenzione provveda a costituire un organismo indipendente e che abbia le condizioni di indipendenza necessarie a permettergli di esercitare efficacemente le funzioni al riparo da ogni indebita influenza. non si tratta di voler sottrarre alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici in generale, il compito di vigilare sulla correttezza dell'operato, che è un obbligo che permane e che ha un suo sbocco nelle eventuali procedure disciplinari, bensì di costituire un'autorità garante della corretta applicazione della Convenzione, che sia indipendente. Effettivamente, l'organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva tutte le caratteristiche di indipendenza, proprio perché inserito nell'ambito del Governo. Per questo con con l'ordine del giorno chiedo la costituzione di una struttura che garantisca le condizioni di indipendenza previste dall'articolo 6. Si chiami Alto Commissario per la corruzione o meno, l'importante è che non sia inserito in una struttura governativa

un organismo quale l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (UNAR), rispetto al quale noi - forse erroneamente - abbiamo resistito

perché prevedeva l'esclusione della possibilità di contestare il delitto di concussione a tutta una serie di persone, indicate all'articolo 322-*bis* del codice penale. faceva riferimento anche a membri del Parlamento europeo, a funzionari e ad agenti assunti all'interno delle Comunità europee a persone comandate.

presso organismi delle Comunità europee - in casi di condanna per delitti quali il peculato, la corruzione, la concussione e reati di tal genere non si applicassero le pene accessorie.

ci trova per metà soddisfatti, nel senso che le pene accessorie sono state reintrodotte nel caso di condanna per i reati di peculato, corruzione e gli altri indicati dagli articoli 316 a 320

proprio nell'ottica suggerita dagli organismi europei. Questi provvedimenti sono stati predisposti da senatori dell'opposizione

nel nostro ordinamento, non si capisce per quale motivo determinate categorie di persone dovrebbero essere escluse dalla punibilità per fatti di tal genere.

*(PD)*. Signor Presidente, il problema della distinzione tra corruzione e concussione si è sempre posto

diventando parte lesa, nell'ipotesi che riuscisse a dimostrare di essere stato concusso, aveva anche diritto alla restituzione delle somme pagate per ottenere i favori che erano stati in effetti ottenuti.

dal fatto tipico che l'autore è un pubblico ufficiale. Si voleva appunto in questo modo cercare di accelerare i processi contro la pubblica amministrazione, ribadendo soprattutto che il fatto grave era che una persona desse soldi a un pubblico ufficiale. Infatti, se non li voleva dare, così come spesso accadeva, poteva non darli semplicemente sporgendo

che agevoli l'amministrazione della giustizia, che renda questi processi più veloci e che punisca con maggior efficacia chi si presta ad ottenere, specialmente negli appalti pubblici, dei privilegi rispetto agli altri, facendo anche nei confronti degli altri una concorrenza sleale, pagando il pubblico ufficiale e cercando un padrino che gli faccia avere con maggiore facilità gli appalti mediante corresponsione di denaro. Propongo, pertanto, e prego il sottosegretario Caliendo di ripensare alla presentazione di un emendamento di questo tipo nel momento in cui si riesaminerà nel suo complesso l'istituto dei reati contro la pubblica amministrazione.

che era perfettamente in linea con i disegni di legge presentati da noi, nel senso che rimaneva il reato di concussione. dal 28 maggio del 2009 ad oggi per cui il Governo ritiene di escludere il reato di concussione per i soggetti che ne possono rispondere, ossia i membri del Parlamento europeo della Corte di giustizia, i funzionari e le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o da soggetto privato? Il soggetto privato comanda presso le Comunità europee un proprio dipendente e, assieme a tutti gli altri soggetti che ho indicato, costui non può rispondere del reato di concussione. Quindi, mentre prima il corruttore diceva di essere stato concusso

preteso denaro abusando del suo ruolo per restare impunito! Ma questa non è né amnistia né indulto! Chi volete proteggere? Non è pensabile che, improvvisamente, venga fuori questa norma! Ci deve essere qualcosa!

caro Sottosegretario. Esisterà quando verrà riformato tutto il capitolo dei reati contro la pubblica amministrazione, quando la concussione diventerà una fattispecie della corruzione con pena adeguata, perché questo noi prevediamo. Oggi la concussione è punita con una pena da 4 a 12 anni; se sparisce se sparisce per alcune categorie di soggetti che possono essere anche privati, che pure svolgono una funzione presso le Comunità europee, non l'avremo per una condotta gravissima, che continua ad essere operante per tanti altri soggetti: avremo una categoria di privilegiati che potranno essere corrotti e diranno di aver costretto alla corruzione, di aver intimorito, il corruttore è una loro vittima. Quindi, festa per tutti! Assolti, non processabili, non imputabili! Ma cosa ci state proponendo! Non è la pena di morte. Voi eliminate un reato per una categoria ristretta di persone e non ve ne rendete conto. Ripeto; eliminato un reato per una categoria ristretta di persone: perché? Perché Perché il funzionario inviato da un soggetto privato a lavorare presso la Commissione europea non può rispondere di concussione e se è lo stesso privato che svolge una funzione di pubblico servizio in Italia invece ne risponde? Ma perché? Perché questa modifica? negli ultimi giorni, perché fino al 28 maggio il Governo aveva proposto un testo che non prevedeva questo. Perché il Governo oggi presenta un emendamento? Ci dica chi protegge!

anche se forse non nei toni eccessivamente accalorati del collega Li Gotti. Ad esempio, nell'ipotesi di reato commesso in concorso

viene processato e condannato per il reato di concussione, mentre il funzionario, il pubblico ufficiale dell'Unione europea no.

è legittimo sospettare - mi sia consentito il termine - che non si vuole ratificare questa Convenzione oppure che la si vuole ratificare solo ed esclusivamente come passaggio formale, affidando poi alla Corte l'ingrato compito di cassare cassare queste disposizioni e, quindi, di vanificarne la utilizzabilità. Ciò rispetto alle cose che qui tutti insieme, maggioranza ed opposizione, abbiamo detto scegliendo di aderire e di ratificare, anche se con ritardo, questa Convenzione.

e le fattispecie così come verrebbero configurate a seguito di questa modifica e dell'entrata in vigore della Convenzione con questa modifica, portano sostanzialmente a trattare condotte illecite identiche in maniera diversa pur, pur, signor Sottosegretario, non essendo in dubbio che la normativa a cui si fa riferimento e che si applica è la normativa italiana, che non può fare distinzione rispetto alla stessa condotta a seconda della qualifica che il soggetto ricopre o della funzione che riveste: questo perché nel nostro Paese non esiste ancora la figura del pubblico ufficiale comunitario distinta dalla funzione del pubblico ufficiale italiano. Questo è il dato. Pertanto, se posso permettermi, insisto perché venga modificata questa disposizione.

perché oggi, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali, il proliferare delle società miste fa sì che molta dell'attività sia sottratta al controllo pubblico, almeno quello che noi intendevamo così. così. Insistere su questo punto significa mettere a serio rischio l'operatività della Convenzione. Fate prima ad assumervi la responsabilità politica di non ratificarla e la chiudiamo qui; ma non facciamo una cosa rispetto alla quale obiettivamente ci rideranno in faccia da tutte le parti del mondo, isole comprese.

non riguarda la concussione nel nostro Paese, ma se nei rapporti internazionali nei confronti di soggetti pubblici ufficiali stranieri

dato tecnico, senza dietrologie politiche che non hanno alcun senso rispetto ad un dato di fatto noto all'opposizione come alla maggioranza e a tutti coloro che, per varie ragioni, hanno avuto occasione di avere rapporti internazionali.

Caliendo da molti anni - tra l'onorare un impegno internazionale ed espungere dal nostro codice il reato di concussione per i parlamentari europei. Cosa c'entra con la possibilità di adeguarsi?

recepimento delle prescrizioni contenute nella Convenzione, nonché l'adeguamento della nostra legislazione nazionale all'impegno sottoscritto da tanti Paesi in ordine ai reati di corruzione (la Convenzione delle Nazioni Unite, firmata nell'ottobre del 2003), cosa c'entra con la nostra legislazione interna, che all'articolo 322-*bis* del codice penale prevede il reato di concussione, tra gli altri, per i membri della Commissione delle Comunità europee del Parlamento europeo, cioè dei parlamentari italiani che vanno in Europa? Lo voglio capire; dalle parole del sottosegretario Caliendo non l'ho compreso

potrei adottare un'espressione utilizzata dal presidente Andreotti: tante volte a pensar male si fa peccato, ma probabilmente ci si prende. Non abbiamo precedenti che ci rassicurino circa un esito negativo dell'indagine di cui parlava il senatore Li Gotti, ma questo lo dovete sapere: state cancellando dal codice penale italiano il delitto di concussione per i parlamentari italiani che vanno a rappresentare il nostro Paese in Europa. Un giorno ci spiegherete anche il perché.

che questo è un emendamento presentato in Aula dal Governo. Sappiamo tutti quanti benissimo che, se si trattasse di emendamenti presentati in precedenza, il termine scadrebbe al momento della discussione generale. In questo caso, l'emendamento è stato presentato in Aula e il primo momento in cui ci viene consentito di chiedere il voto segreto Quindi, credo si presenti una fattispecie nuova rispetto a situazioni precedenti.

La seduta è ripresa. La Presidenza è venuta a conoscenza che i Capigruppo hanno trovato la soluzione. Per avere nella disponibilità il documento che è stato sottoscritto, sospendo la seduta per altri dieci minuti.

La seduta è ripresa. è stato presentato l'ordine del giorno G3.100, a firma dei capigruppo Gasparri, Bricolo, Finocchiaro, D'Alia, Pistorio e Belisario. Invito il senatore Segretario a darne

considerata la necessità di adeguare l'ordinamento italiano alla Convenzione OCSE del 1997 sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri; vista la raccomandazione dell'OCSE con cui si invita il Governo italiano ad escludere la configurabilità dal reato di concussione rispetto al reato di corruzione dei pubblici ufficiali stranieri; atteso il comune impegno di tutti i Gruppi a pervenire mediante le vie regolamentari più rapide alla riforma della materia in applicazione delle convenzioni internazionali, impegna il Governo a ritirare l'emendamento 3.100 (testo 2)».

tra tutti i Gruppi, si è convenuto che la proposta del Governo non intende dare benefici di impunità a chicchessia, né italiano né straniero, ma semplicemente ottemperare a quell'invito che è venuto da organismi internazionali, l'OCSE ed altri, affinché l'ordinamento italiano non lasci margini di ambiguità dovuti a una specificità del nostro ordinamento, che accanto al reato di corruzione prevede anche il reato di concussione. Altre legislazioni non prevedono questa fattispecie e da qui l'orientamento, la sollecitazione, il richiamo al Governo italiano a chiarire la normativa, in particolare per gli stranieri che operano in Italia; quindi nessuna forma di impunità per nessuno. Atteso che questo è l'obiettivo condivisibile del Governo, che tra l'altro non può che attivarsi per rispettare una sollecitazione che invita l'Italia a uniformarsi a convenzioni internazionali che risalgono addirittura gli anni '90, l'ordine del giorno G3.100 che abbiamo concordato, con una formula originale, ma di chiaro significato politico, invita il Governo a ritirare l'emendamento 3.100 (testo 2), ma nella premessa c'è la chiara affermazione di volontà del Senato - tutto il Senato, con la firma di tutti i Capigruppo - di procedere, nelle forme più rapide che il Regolamento consentirà, a partire dalla Commissione giustizia, ad approvare una normativa che sia in linea con i richiami internazionali che puntano a una omogeneità dell'impianto penale e sanzionatorio e a non creare sacche di impunità. C'è stato un chiarimento che per quanto riguarda il nostro Gruppo è ampiamente soddisfacente. Voglio ringraziare il sottosegretario Caliendo per la collaborazione giuridica oltre che istituzionale, come membro del Governo, e anche i colleghi Capigruppo perché siamo riusciti a trovare una volontà unanime di garantire il rispetto di convenzioni internazionali nella chiarezza dell'impianto sanzionatorio. Per questo motivo sosteniamo con convinzione l'ordine del giorno G3.100 e l'attività legislativa che già dai prossimi giorni, sulla base di testi esistenti o delle proposte che sorgeranno, possa rapidamente consentire alla Repubblica italiana di adempiere a obblighi internazionali. Presidente, vorrei esprimere soddisfazione rispetto alla soluzione che abbiamo trovato, e che ci pare la più adeguata dinanzi alla delicatezza della questione. ovviamente resiste ed è interesse comune - non soltanto del Governo e della maggioranza, ma anche dell'opposizione - la ratifica della Convenzione, l'emendamento del Governo, di fatto, lasciava scoperta una condotta che oggi, nel nostro codice penale, all'articolo 322-*bis*, qualifichiamo come corruzione riconducibile a parlamentari europei, membri della Commissione e via dicendo. Residuava quindi un comportamento che però, a norma del nostro sistema penale, così come modificato con l'emendamento del Governo, non poteva essere sussunto in una fattispecie tipica.

ragionevole. In Commissione esteri, in seduta congiunta con la Commissione giustizia, stiamo già lavorando alla rimodulazione dei reati contro la pubblica amministrazione, con la sparizione del reato di concussione che diventa una particolare condotta del reato di corruzione. Questo è il nostro obiettivo, perché la concussione escludeva una condotta illecita, ossia quella del corruttore. L'Europa, attraverso i suggerimenti che ci sono pervenuti da parte dell'OCSE, voleva estendere il presidio penale su alcune condotte. Ciò che stavamo attuando andava in senso contrario. Ora lavoreremo in questa direzione e siamo già in fase avanzata di

su alcune condotte illecite, eliminando un reato che sta diventando anacronistico, essendo divenuto lo strumento per escludere la responsabilità del corruttore. In questa direzione condividiamo il lavoro che è stato svolto d'intesa da tutti i Gruppi e con soddisfazione prendiamo atto anche della enuncianda adesione del Governo alla nostra sollecitazione.

che vanno tutte nella stessa direzione. Non vi è contrapposizione rispetto al merito delle questioni quando si affrontano con responsabilità. L'impegno da parte del nostro Gruppo è eventualmente teso

accetta di ritirare l'emendamento, tenendo conto dell'impegno dei Gruppi parlamentari ad affrontare la questione. Non voglio

la lotta alla corruzione. Si tratta di un fenomeno di vastità elevata anche a livello mondiale, che minaccia la stabilità e la sicurezza delle società danneggiandole anche da un punto di vista economico-finanziario, ed ha per dichiarato oggetto un punto che noi del Gruppo parlamentare UDC-SVP-Autonomie riteniamo molto importante: la promozione, il sostegno e la facilitazione della cooperazione internazionale e della relativa assistenza tecnica ed amministrativa ai fini della prevenzione di fatti di corruzione e di recupero dei proventi del reato.

fortemente atteso; si tratta ora - a mano a mano arriveranno anche gli altri - di ratificare tutte le Convenzioni che noi abbiamo già firmato e che da alcuni anni aspettano di essere ratificate dal nostro Paese. Questo è un altro tassello che va nella direzione della lotta contro la corruzione per l'affermazione di un'economia pulita, che veda i cittadini uguali nel mercato e nel rispetto delle regole. Il nostro voto, pertanto,

Nel novembre 2006 il Parlamento europeo aveva sollecitato gli Stati membri ad aderire e a ratificare senza ulteriori ritardi questa Convenzione. Noi lo facciamo oggi, in una giornata particolarmente importante perché questa mattina abbiamo votato l'adesione del nostro Paese al Trattato di Prum per la cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina;

con i necessari adeguamenti della legislazione nazionale. Si tratta di un atto di assoluto rilievo, sia nazionale che internazionale, perché interviene in un settore della vita sociale, politica ed economica particolarmente sensibile. Questo è il primo accordo che interviene a livello mondiale in tema di prevenzione e di contrasto alla corruzione come fenomeno sovranazionale, che attraversa trasversalmente tutti i Paesi del mondo e tutti i regimi. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e la stessa Banca mondiale, partendo da analisi e dati approfonditi e particolareggiati, lanciano un preoccupato allarme sui rischi determinati a livello di rapporti internazionali dal fenomeno della corruzione. fenomeno mette seriamente a rischio la stabilità e la sicurezza delle società, costituendo un freno consistente allo sviluppo dell'economia e ai rapporti economici e finanziari corretti e trasparenti. trasparenti. In particolare, rompendo gli schemi della legalità e facendo strame delle regole, esso danneggia i settori ed i soggetti più deboli della società, creando un *humus* particolarmente fertile per lo sviluppo della criminalità, anche organizzata, e al contempo divenendo strumento per la degenerazione del tessuto sociale

Anzi, i dati statistici, europei e mondiali, collocano il nostro Stato e le nostre amministrazioni ad un livello di corruttela non degno di un Paese civile. Forse non è solamente un caso se attendiamo la ratifica di questa Convenzione ONU da circa sette anni e se, anche questa volta, l'Italia si pone in coda all'elenco degli Stati che hanno già provveduto, in larghissima parte, alla ratifica. È ovviamente con soddisfazione che rileviamo come l'iniziativa legislativa anche in questa XVI legislatura sia nostra, del Partito Democratico *in primis*, così come dei colleghi dell'Italia dei Valori, mentre il Governo, che inizialmente richiedeva continui rinvii si sia alla fine accodato alla nostra iniziativa. Peraltro, va dato atto che alla redazione del testo presentato oggi testo presentato oggi hanno partecipato fattivamente e positivamente, all'interno di un apposito Comitato ristretto, i senatori della 2a e della 3a Commissione, sia di maggioranza che di opposizione. In conclusione, come gruppo del Partito Democratico, riteniamo che il disegno di legge in esame fornirà alle forze di polizia e alla magistratura, nell'ambito delle diversificate competenze nazionali, maggiori e più efficaci strumenti in materia di prevenzione e di contrasto alla corruzione, aumentando gli spazi della cooperazione internazionale, ampliando i mezzi di assistenza tecnica, rendendo più efficaci le attività rivolte in particolare al recupero e alla confisca dei beni, promuovendo sistemi volti a garantire trasparenza e buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. Per questo motivo, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del

il parere è contrario. Posso comunque assicurare i firmatari dell'ordine del giorno e l'Aula che il primo punto del dispositivo è all'attenzione prioritaria del Governo, il quale ha la ferma intenzione di provvedere, appena possibile, al rifinanziamento

e rifinanziare urgentemente il Fondo per lo sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, per poter assolvere agli impegni previsti dalle Convenzioni di Ottawa e di Oslo a cui l'Italia ha aderito.

- dice che: «possono essere oggetto di scambio diretto tra i due Paesi contraenti o anche tra aziende private autorizzate diverse tipologie di armi, tra le quali anche le mine e i loro dispositivi di controllo», senza alcuna specificazione sul tipo di mina.

Stiamo parlando di mine antiuomo; vi invito solo a riflettere. Se due mesi fa avete fatto un errore lo sapremo oggi con questo voto, ma quel rosso (ve lo ripeto con il cuore da padre

riguardano i diritti umani. Invito i colleghi a riflettere sull'articolo 5. Lo faccio perché sono cosciente,

volevo semplicemente ricordare al collega Pedica che esistono due tipi di mine, le mine antiuomo e le mine anticarro. Ora, io credo che dal punto di vista semantico la differenza tra un carro e un uomo sia conosciuta persino a lei, senatore, quando noi votiamo lo scambio di mine, evidentemente sono mine solo anticarro, proprio perché abbiamo votato a larga maggioranza un embargo sulle mine antiuomo. Stia tranquillo, non è sangue. Casomai sarà soltanto l'olio che uscirà dai carri dei nemici che si alzeranno in aria. Oddio, con qualcuno dentro, ma pazienza!

il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007

ha volontà di rafforzare i legami e gli scambi culturali con l'Italia, particolarmente nel settore dell'istruzione. È soprattutto un Paese cardine nell'equilibrio mediorientale. Come tutti sappiamo, fin dal 2002

con il riconoscimento dello Stato palestinese e con una giusta soluzione per i rifugiati. Quindi, sappiamo tutti che si tratta di uno Stato veramente chiave negli equilibri mondiali e negli equilibri della regione mediorientale. Premetto questo perché mi sembra importante ricordarlo.

a riferire puntualmente, ove ritenuto necessario ed opportuno, sulla materia oggetto dell'Accordo e sugli scenari internazionali nel cui ambito quest'ultimo opera.

di una gravità estrema, risiede nell'articolo 7 in cui si prevede una clausola di rinnovo automatico dell'Accordo ogni cinque anni, a meno che uno dei due Paesi non comunichi anticipatamente, sei mesi prima del rinnovo, di non voler procedere in tal senso. Data l'estrema fluidità politica dell'area mediorientale e la concreta possibilità di capovolgimenti degli equilibri interni all'Arabia Saudita, rinnovare di ulteriori cinque anni un impegno così importante e sensibile per l'Italia, come quello nel settore della difesa (che prevede scambio di materiali bellici, addestramento congiunto e scambio di informazioni militari), appare inadatto un rinnovo del tipo silenzio-assenso. Pertanto, con l'ordine del giorno G100 si chiede che, almeno 9 mesi prima del tacito rinnovo il Governo consulti le Camere attraverso il dibattito ed il voto parlamentare per decidere se le condizioni interne al Paese saudita nonché la geopolitica regionale dell'area mediorientale

del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma

Ma fin qui si tratta di valutazioni politiche relativamente al proibizionismo a livello mondiale in materia di sostanze stupefacenti. Quello che però credo vada ricordato è che per questi crimini in Arabia Saudita vige la legge del taglione e anche la pena di morte. Tra l'altro, dopodomani è la Giornata mondiale contro le droghe che, cinque o sei anni fa, grazie alla gestione del neo eurodeputato dell'Italia dei Valori Pino Arlacchi, si festeggiava con impiccagioni pubbliche tanto in Cina, quanto in Iran, quanto in Arabia Saudita. Siccome andiamo a firmare un Trattato bilaterale in materia di controllo della criminalità organizzata e siccome all'articolo 5 di questo Accordo bilaterale si prevede che in alcuni casi entrambe le parti contraenti possono rifiutare completamente o parzialmente la cooperazione, se questa è in conflitto, tra le altre cose, con la normativa nazionale, oppure se è in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio, che cosa potrebbe succedere ad un cittadino italiano o dell'Unione europea colto nell'atto di comprare, spacciare o consumare sostanze stupefacenti come arbitrariamente catalogate nella Convenzione del 1988? Ci potrebbe essere il rischio della pena di morte. Allora, visto e considerato che il nostro Paese invece nel mondo è noto per la campagna per la moratoria universale della pena di morte, chiediamo al Governo di impegnarsi a monitorare costantemente l'applicazione dell'Accordo al fine di garantire che le norme codificate negli strumenti internazionali dei diritti umani, ratificate dall'Italia, siano rispettate pienamente in ogni circostanza. il regno monarchia assoluta non costituzionale di valore teocratico Arabia Saudita non ha ratificato nessuno degli strumenti internazionali che garantiscono i diritti umani fondamentali. Quindi, per ottenere il voto favorevole che altrimenti sarebbe di astensione della delegazione radicale, ma penso di tutti coloro i quali hanno a cuore - e ce ne sono molti qui dentro - il valore e la tutela dei diritti umani, come minima riduzione di quello che potrebbe essere un danno (e nelle carceri dei Paesi arabi ci sono molti italiani che vi restano per motivi di traffico di sostanze stupefacenti), almeno un parere favorevole e quindi l'impegno assunto da parte del Governo relativamente al monitoraggio costante dei diritti umani potrebbe rappresentare un minimo passo nella direzione giusta.

Il Governo comprende in pieno lo spirito dell'ordine del giorno e agisce con convinzione in tutti i fori multilaterali per la tutela e la promozione dei diritti umani, con particolare riguardo alla battaglia per la moratoria e l'abolizione della pena di morte. Infatti, in questo ambito, di concerto con i partner europei, si può efficacemente monitorare il rispetto delle norme e degli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le Istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri

o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione europea di gestione delle crisi. Esso è finalizzato ad

che la ratifica del Trattato rappresenti un ulteriore ed importante slancio del nostro Paese verso il percorso di collaborazione europea, il cosiddetto secondo pilastro.

Sono stati arrestati 25 giornalisti e 500 uomini vestiti di nero e armati di mazze hanno ferito gravemente ed ucciso delle donne fuori da una moschea.

Presidente, quello che sta accadendo in Iran in questo momento purtroppo era largamente prevedibile. Gli atteggiamenti che il Governo di quel Paese ha posto in essere in questi giorni facevano presentire un'*escalation* della violenza, ed è la ragione per la quale senatori di ogni schieramento di ogni schieramento politico di quest'Aula, anche in modo silenzioso, avevano manifestato, nei giorni scorsi, simbolicamente la loro preoccupazione ed il loro apprezzamento nei confronti del modo non violento in cui

al Governo di venire a riferire prontamente non solo su quello che sta accadendo, ma anche su quali passi, assai più vigorosi e forti di quelli sin qui posti in essere, il Governo italiano intende fare, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, per fermare questo eccidio insopportabile. *(Applausi

attenzione alla democrazia che c'è in altri Paesi, se poi qui non riusciamo neanche a stare minimamente attenti, dopo aver richiamato la pericolosità di alcuni Governi nei confronti della

dalle teocrazie islamiche, dovevano far capire la pericolosità di certi Stati e di certi dittatori, senza aspettare questi eventi. Il fatto che in Italia

sta ulteriormente a significare da che parte sta l'Italia: sicuramente, non dalla parte delle teocrazie poco responsabili e poco democratiche verso i loro popoli. Presidente, colleghi, il momento particolare ci obbliga ad evitare di pronunciare dichiarazioni di parte. Ci troviamo di fronte ad una tragedia annunciata,

G8, ritengo che il Parlamento e certamente il Governo abbiano la necessità di far sentire, in modo chiaro e forte, l'imbarazzo e lo sdegno. Quando le manifestazioni di piazza, anche le più vivaci, sfociano in una repressione sanguinosa, questo allarma le coscienze, mortifica la democrazia, ci spinge a richiedere un anelito di libertà sempre più marcato e sempre più forte, perché questa è la base dello sviluppo dei Paesi moderni. Chiediamo che il Governo anticipi il suo intervento alle Commissioni congiunte, perché tutto nasce da un'incertezza di fondo sulle libere, tra virgolette, elezioni che ci sono state nei giorni scorsi nella Repubblica islamica dell'Iran. Chiediamo che tutti gli organismi internazionali, a cominciare dall'ONU, intervengano senza voler mettere il naso nelle cosiddette democrazie islamiche, ma mettendoci le mani, perché abbiamo la preoccupazione che quelle elezioni possano segnare l'inizio di un massacro barbaro degli oppositori.

Volevo solo precisare che, come ha detto la Presidente, il ministro Frattini dovrebbe venire mercoledì a riferire alle Commissioni esteri di Camera e Senato. Domani il ministro Frattini è a Trieste, impegnato per il G8. Questa era l'informazione che avevamo prima di questi tragici avvenimenti. Capiamo perfettamente che a Trieste comincia il e chiedo al Governo - se non sia il caso, alla luce degli avvenimenti di cui abbiamo notizia, che invece la relazione al Parlamento avvenga in date più ravvicinate.

Signora Presidente, mi associo, a nome del Gruppo del Partito Democratico, alla sua sollecitazione al Governo. Il Ministro degli affari esteri, poco fa, ha definito orribili i fatti che stanno accadendo a Teheran. Il Senato si è espresso con una condanna unanime, tutti i Gruppi hanno espresso lo stesso giudizio. Credo che sia una situazione di una gravità estrema e che aspettare una settimana sia assolutamente non ammissibile. Quindi, chiedo al Sottosegretario di pregare il Ministro di fare in Parlamento, domani mattina, una relazione su quello che sta accadendo a Teheran e sulle iniziative del Governo italiano.

alle Camere sui fatti tragici di Teheran, ma che sia anche necessaria ed urgente un'immediata iniziativa diplomatica del Governo, con un richiamo all'ambasciatore iraniano in Italia, perché credo che la situazione che si vive in quel Paese sia di estrema gravità e noi dobbiamo fare sentire con i fatti la condanna del nostro Paese, anche in ragione dell'incontro del G8 dei prossimi giorni.

già questa sera emettere un comunicato in cui esprimiamo la nostra critica e il nostro sdegno, dal momento che siamo autorizzati a farlo. Perché attendere che il Governo venga a riferire? I fatti sono chiari: ascolteremo il Governo e discuteremo della politica internazionale, ma mi chiedo perché il Senato della Repubblica non debba esprimere in poche righe, autonomamente e immediatamente, il proprio sdegno per quello che sta accadendo.

la difficoltà del settore agroalimentare stia oggi attanagliando molte imprese. Stiamo parlando di una preoccupazione

quale debba essere l'azione straordinaria e assolutamente eccezionale del Governo se vuole rendere centrale la questione agroalimentare. Sono quattro i punti da affrontare sull'emergenza: vi è il tema del credito e dell'indebitamento delle imprese;

il rifinanziamento del fondo di solidarietà

è l'urgenza di una rinegoziazione dei mutui di chi ha investito in questi anni e non riesce ora a far fronte alla restituzione. Abbiamo urgenza di affrontare la questione della dilazione delle rate e dell'abbattimento dei tassi che oggi sono ancora più alti che in altri settori. Sono misure da richiedere e attuare immediatamente.

alla ristrutturazione del settore. Servono misure urgenti per la concentrazione dell'offerta agricola, un rafforzamento del dimensionamento o delle forme di aggregazione. subito aiuti straordinari per l'internazionalizzazione della rete distributiva del comparto perché il settore agroalimentare italiano, caratterizzato da tipicità e valori territoriali, possa accelerare l'inserimento nei mercati esteri; quando parliamo di internazionalizzazione, non intendiamo solo l'*export*, ma una presenza consolidata e duratura nei Paesi extraeuropei, nuove *partnership* commerciali e nuove relazioni bilaterali. Chiediamo aiuti straordinari ed incentivi

di ristrutturare e riconvertire le filiere particolarmente toccate della crisi economica generale, cui si sono sovrapposte le politiche europee che sono state particolarmente penalizzanti per questi settori. Chiediamo, dunque, che il Governo avvii davvero un'inversione di tendenza. In un anno, a differenza di altri Paesi come la Francia (che ha investito 250 milioni di euro per far ripartire il settore, per difendere e sostenere i redditi degli imprenditori agricoli),

Credo occorra in particolare sostenere quella impresa agricola che assicura al nostro Paese forza economica ed occupazione stabili, presidio ambientale, sicurezza alimentare e soprattutto promuove l'immagine di un Paese laborioso, in grado di conquistare i mercati mondiali con i prodotti di grande qualità, cioè quelli del *made in Italy*.

onorevoli colleghi, nell'ambito del dibattito sulle mozioni sulla crisi del settore agroalimentare, con particolare riferimento alle politiche che il Governo dovrà adottare per aumentare la competitività del comparto, vorrei esprimere un apprezzamento sulla mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico, nei confronti della quale non possiamo che esprimere un voto favorevole. Peraltro, tutti i temi trattati nella mozione dei colleghi del Partito Democratico, ampiamente condivisi dal Gruppo dell'Italia dei Valori, sono sempre stati sostenuti con forza e convinzione anche in sede parlamentare e, in particolare, nell'ambito della Commissione agricoltura anche nel corso delle audizioni svolte con le organizzazioni professionali, produttive e sindacali del settore, laddove abbiamo sempre condiviso il forte disagio che sta colpendo il comparto agroalimentare e della pesca. Pertanto, riteniamo che gli impegni richiesti al Governo nella mozione n. 85 (testo 2) siano puntuali ed efficaci e, ove accolti e compiutamente realizzati dall'Esecutivo - in verità molto distratto, se non addirittura sordo, ai richiami del mondo agricolo italiano possano offrire all'intero comparto del settore agroalimentare e della pesca una preziosa opportunità di crescita, così come risulta necessario soprattutto in un momento in cui gli elementi di debolezza del settore sono amplificati dalla crisi congiunturale in atto con la conseguente volatilità dei prezzi e l'estrema difficoltà di accesso al credito da parte degli operatori del settore. Tuttavia, colleghi, nella mozione n. 85 (testo che riguarda i contenuti in merito alla questione meridionale. Noi del Gruppo dell'Italia dei Valori abbiamo voluto quindi presentare una mozione sui medesimi temi del sostegno alla competitività del settore agroalimentare, puntando tuttavia alla necessità di intervenire con maggiore forza e convinzione nei confronti delle aziende agricole del Mezzogiorno. Ciò risulta oggi tanto più urgente in quanto, come emerge dai dati dei maggiori istituti di analisi e di studio, con particolare riferimento a quelli diffusi dal Rapporto Svimez 2009, si conferma che l'economia del Mezzogiorno, da sette anni consecutivi ormai, cresce meno del Centro Nord: nel 2008 il Mezzogiorno ha segnato rispetto all'anno precedente un calo di PIL cento, risultato lievemente peggiore del Centro Nord. Negli otto anni esaminati dallo Svimez, che vanno dal 2000 al 2008, appare evidente che il Sud è cresciuto meno della metà del Centro Nord, nonostante l'utilizzo dei fondi strutturali. Questo è un dato preoccupante: nonostante le ingenti risorse, la qualità della spesa dei fondi comunitari delle Regioni meridionali non ha determinato alcun incremento del PIL e, dunque, alcuna crescita socio-economica del territorio. La crisi del Mezzogiorno è la crisi del sistema Paese Italia, per far fronte alla quale occorre una assunzione di responsabilità da parte del Governo per trasformare l'attuale crisi in opportunità e per rilanciare politiche industriali che garantiscano lo sviluppo equilibrato del Paese e non penalizzino il Sud. È evidente che, se si intende avviare tale processo strutturale, non si può continuare a saccheggiare le risorse FAS. Il Mezzogiorno e l'agricoltura meridionale nel suo contesto, hanno bisogno di una terapia d'urto per avviare un'inversione di tendenza che certo non si costruisce dall'oggi al domani, ma che è colpevole rimandare ancora. Dal Rapporto Svimez 2009 emerge la costante del dualismo Nord Sud, con un Meridione che esprime timidi segnali di ripresa (ma inferiori ad altre aree deboli dell'Unione europea e, comunque, non in agricoltura). Il sistema agricolo del Mezzogiorno sta perdendo competitività e permangono forti divari strutturali ed organizzativi per il sistema delle imprese con il resto dell'Italia e dell'Unione europea. Il settore agricolo e agroindustriale è da sempre nel mirino strategico comunitario, che con la programmazione dei fondi 2007-2013 affida al Mezzogiorno un posto di primo piano in tema di aiuti per lo sviluppo rurale. In linea con i dettati comunitari, anche i documenti programmatici regionali italiani devono sostenere un modello di sviluppo ancor meglio integrato, che non soltanto valorizzi le precedenti esperienze ma assegni una moderna centralità alle aree interessate da produzioni agricole, favorendo l'idea di una nuova e rinnovata ruralità e del modello europeo di agricoltura.

tornare tutti quanti a casa. Se abbiamo deciso di tornare a casa evitando di parlare e di pensare che c'è gente che soffre in questo settore significa che non c'è la responsabilità da parte dei colleghi di voler ascoltare. *(Commenti

corretto) intendiamo discutere e portare all'attenzione dell'Aula il problema della salvaguardia del sistema agroalimentare italiano e delle sue produzioni di qualità, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo e del ministro Zaia a cui il mio Gruppo è particolarmente sensibile ed attento.

particolare ne elenco cinque: gli ammortizzatori sociali, necessari per governare la crisi che sta interessando le imprese del settore; il sistema assicurativo e il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale;

sulle misure relative agli aiuti di Stato alle imprese, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, che costituisce il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi Per quanto concerne gli aspetti attinenti all'attuazione dei meccanismi di gestione del rischio in agricoltura, si ritiene opportuno segnalare il regime di aiuti di Stato n. XA 396/08 che prevede la concessione di contributi per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili e altre calamità e perdite dovute a epizozie e fitopatie. In merito agli incentivi assicurativi, occorre premettere che lo stanziamento recato dalla legge finanziaria 2008 è stato di 220 milioni di euro; a seguito della decurtazione di 32 milioni di euro

Per il pagamento dei saldi contributivi del 2008, è intervenuta a fine anno una ulteriore disponibilità di 66 milioni di euro, grazie ad un emendamento all'articolo 1-*bis* della legge 30 dicembre 2008, Con le attuali disponibilità, è possibile assicurare l'erogazione del contributo nella misura del 47 per cento. Per il 2009, invece, la legge finanziaria non ha previsto uno stanziamento specifico; considerando una base assicurativa nel limite del 2008, incrementata di fabbisogno di spesa sarà di circa 230-240 milioni. Occorre, pertanto, assicurare un'adeguata copertura a tale intervento anche perché gli strumenti comunitari recentemente attivati nel quadro della *health check* non potranno entrare in funzione prima del 2010. agricole, alimentari e forestali, nell'ambito degli obiettivi operativi concernenti la promozione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura e promozione della formazione professionale dei giovani agricoltori, ha ha disposto: la concessione di borse di studio per frequenza di *master* universitari, ovvero organizzazione attraverso istituti specializzati di *master* di formazione imprenditoriale in agricoltura; l'erogazione di premi e contributi per la partecipazione a concorsi, *forum* e fiere alle aziende agricole condotte da giovani che si sono distinte per l'innovazione dell'esperienza l'erogazione di contributi per progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo proposti da piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori con la collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca; l'erogazione di contributi per la sostituzione di giovani imprenditori in caso di malattia, infortunio, maternità o frequenza di corsi di formazione. Attraverso l'Osservatorio per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile sono inoltre allo studio proposte di finanziamento di misure per l'agevolazione dell'accesso al credito da parte dei giovani imprenditori e ciò in linea anche con quanto sollecitato nelle mozioni parlamentari in oggetto. Le risorse necessarie ad attuare le citate iniziative derivano dal «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», istituito con la legge n. 296 del 2006, che stanziava 10 milioni di euro l'anno per 5 anni a partire dal 2007. Si evidenzia tuttavia che a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di legge in materia economica, la dotazione finanziaria a disposizione del Ministero per gli interventi sopra descritti si è ridotta a 5 milioni di euro. Per quanto sopra esposto si evidenzia che l'azione di questo Ministero in questa particolare area d'intervento è rivolta a quei giovani imprenditori agricoli che già esercitano l'attività e sono titolari d'impresa, mentre il maggior impegno richiesto attraverso la mozione in argomento appare indirizzato, pur nelle attuali difficoltà economico-finanziarie, a creare nuove opportunità per «attrarre e motivare l'ingresso di giovani figure imprenditoriali» nel settore agroalimentare e della pesca.

In ordine al problema delle contraffazioni, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero sta lavorando in sede nazionale ed internazionale per migliorare le norme legate ai prodotti di qualità,

Presidente, colleghi, come accade per tutti i settori dell'economia a livello mondiale ed italiano, anche quello agricolo del nostro Paese risente del particolare momento di recessione economica.

Ci accorgiamo che l'agricoltura, l'*export* agricolo sta perdendo terreno, ma ne sta perdendo meno, molto meno, di altri settori della nostra economia. Bisogna lavorare sul controllo dei prezzi al consumo continuando a portare avanti iniziative che promuovano i mercati agricoli con le vendite dirette degli agricoltori. Dobbiamo continuare a sostenere il Governo nelle importanti e innovative iniziative riguardanti la tracciabilità e l'etichettatura, dando un documento, una sorta di carta di identità, ai nostri prodotti,

un disegno di legge relativo proprio alla dieta mediterranea nelle scuole e nelle mense pubbliche. Vanno combattute ancora più efficacemente tutte le forme di contraffazione dei prodotti che, oltre a fuorviare i nostri consumatori, possono creare un grave danno alla salute dei cittadini. Certo, i nostri agricoltori vanno aiutati, sostenuti, soprattutto in questo momento momento di particolare difficoltà, con un'apertura del sistema creditizio per affrontare gli impegni a breve termine, ma dobbiamo intervenire anche con iniziative finalizzate a favorire interventi sul parco macchine del mondo agricolo. interventi quali la rottamazione e incentivi economici all'acquisto di nuovi prodotti possibilmente alimentati con fonti energetiche alternative ed ecocompatibili. Anche la Comunità europea ha recentemente pubblicato una comunicazione a sostegno dell'accesso al finanziamento per consentire agli Stati membri di intervenire a favore dell'agricoltura.

in essere. La difesa del *made in Italy* agroalimentare passa attraverso la cosiddetta tolleranza zero. Occorre dare certezze non solo agli imprenditori agricoli particolare a quelli del Nord Italia, ma anche e soprattutto al consumatore, sempre più esigente e desideroso del rispetto del suo diritto di scelta. L'economia e le imprese agricole alimentari sono sottoposte, al pari di di ciò che sta accadendo al sistema economico nazionale, in modo diretto e indiretto alle conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale, i cui segnali sono ben manifesti. Dobbiamo essere uniti, fatto che la vera sfida non è tra di noi o tra le compagini politiche, ma che la vera sfida è la globalizzazione. I veri nemici sono i prodotti a costi bassissimi, i prodotti contraffatti

Signora Presidente, vorrei far notare all'Aula e a lei che il parere su queste mozioni è stato dato dal Sottosegretario alla giustizia. Ciò dimostra quanta attenzione vi sia, da parte del Governo, nei confronti del settore agricoltura e agroalimentare. Evidentemente il ministro Zaia e il sottosegretario Buonfiglio avevano ben altro da fare

maggioranza. In un momento in cui riflessi della pesante crisi congiunturale che attraversa il Paese gravano sempre più pesantemente su questo settore, la collega Pignedoli ha presentato, nella mozione, una serie di proposte di misure straordinarie. di proposte di misure straordinarie. Da una parte si consentiva una tipologia di intervento, e cioè misure immediate, per la tenuta competitiva del settore. Ci riferiamo all'attivazione di tutti gli ammortizzatori sociali per le imprese agricole agricole e il settore ittico, alla conferma biennale degli sgravi contributivi, alla stabilità fiscale per gli agricoltori, al rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale e, infine, all'incentivazione per l'imprenditoria femminile e giovanile. Ma proponevamo anche un altro sistema di intervento, più strutturale, che serviva a garantire l'intero rilancio del settore, come la concentrazione dell'offerta produttiva per eliminare il triste fenomeno della frammentazione delle nostre imprese agricole, imprese agricole, l'incentivazione ai giovani e alle donne che volevano cimentarsi in questo settore, dato che ormai le nostre imprese agricole scontano un'età che si avvicina intorno ai sessant'anni, e, infine, interventi per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, la difesa dell'origine e soprattutto del *made in Italy*. Quando ho fatto la battuta iniziale, volevo solo ricordare a noi tutti che abbiamo votato qui tre provvedimenti che hanno riguardato l'agricoltura: il decreto-legge anticrisi, in cui la parola «agricoltura» non compariva in alcun modo; il disegno di legge di conversione del decreto sulla competitività del settore agroalimentare,

parlamentari di tutti i colleghi, anche per l'incoerenza degli stessi proponenti che proprio in questi giorni, a causa delle avverse condizioni climatiche, hanno presentato interrogazioni al Governo - e mi riferisco anche ai membri di questa maggioranza - per chiedere il rifinanziamento del fondo Ancora, ricordo il tema della sicurezza alimentare, in merito al quale siamo tuttora in attesa di una risposta chiara, al di là dei pronunciamenti relativi alla contraffazione, sull'avvio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.

ha ritirato il disegno di legge, non spiegandone in alcun modo il motivo. Ovviamente vi è un braccio di ferro all'interno della maggioranza, perché abbiamo saputo lo stesso giorno che è stato presentato alla Camera un decreto-legge con la firma di Zaia sullo stesso tema, quello dell'etichettatura sui prodotti alimentari. Penso che è ora di finirla con questi balletti. Ecco perché finiamo sempre ad ora tarda a parlare di questi argomenti: evidentemente crea qualche imbarazzo

né gli agricoltori né i consumatori e la smetta di andare in qualunque convegno a preannunciare questo disegno di legge. Come Partito Democratico sono stanca di dire che siamo pronti a votare una legge. Tra l'altro, noi stessi abbiamo votato la scorsa legislatura la legge sull'etichettatura dell'olio

ad altri settori, crisi alla quale non si possono dare risposte superficiali o dettate dall'opportunismo. Questo è stato il motivo che ha indotto il Partito Democratico a presentare una serie di proposte

motivo sosterremo la nostra mozione. Al mio intervento saranno allegati gli interventi della collega Antezza e del collega Andria. Però voglio solo dire che ancora una volta questo Governo si mostra assente e questo settore purtroppo non è presente nell'agenda politica del Governo di centrodestra e del Governo nordista di Berlusconi e Zaia.

illustri colleghi, devo notare con un po' di dispiacere che al secondo settore economico del Paese, qual è l'agricoltura, non sempre viene dedicata in termini di tempo l'attenzione che meriterebbe. Voglio ricordare che dopo il settore metalmeccanico, il sistema agroalimentare del nostro Paese, Paese, il più importante d'Europa per il valore aggiunto e secondo - se la batte con la Francia - per quanto riguarda il fatturato, attribuisce al nostro PIL un valore che alcuni stimano superiore ai 220 miliardi di euro, secondo qualcuno addirittura 240. Ma, come sapete, le statistiche sono un po' ballerine.

Semmai ho sempre visto una volontà comune alla collaborazione, a venirci incontro con attenzione, nonché il rispetto e la comune valutazione che l'agricoltura è importante in un Paese industriale e post‑industriale come il nostro. Non è affatto vero che l'agricoltura è un settore residuale. È certamente un settore in crisi, ma non più di altri. A questo riguardo, voglio dire che

dell'opposizione), giacché recita testualmente che il Governo si è contraddistinto esclusivamente per i vistosi tagli a sfavore del comparto agroalimentare. Voglio ricordare che il presidente Berlusconi, il ministro Zaia, ed il Governo nel suo complesso, hanno dovuto in quest'anno dedicarsi alla soluzione di molti problemi che da troppo tempo non erano stati risolti. Sotto il profilo fiscale è stato superato il problema che era stato creato dal Governo precedente in materia di ICI dei fabbricati rurali

la questione dell'IRAP, quest'ultima molto attesa dagli agricoltori. È stata anche risolta fino alla fine di questo anno la questione importante per l'agricoltura del Mezzogiorno - collega di Nardo, lei lo sa perfettamente come me - delle agevolazioni contributive; inoltre risolta dal ministro Sacconi la questione dei *voucher* per i lavoratori a tempo determinato. Onestamente è un po' difficile dire che questo Governo si è disinteressato dell'agricoltura.

un pieno riconoscimento di quanto il Governo sta già facendo. Ad esempio, in merito al fondo di solidarietà nazionale, lei, senatrice Mongiello, sa perfettamente che lo stesso Presidente del Consiglio in prima persona si è recentemente impegnato a trovare le risorse finanziarie sufficienti a dare mandato al ministro Zaia per poter operare di conseguenza. La nostra mozione è stata illustrata in maniera perfetta, come sempre, dal nostro capogruppo in Commissione,

di ritornare al più presto a parlare di agricoltura e di sistema agroalimentare in questa Aula. Credo non sia il caso di ritagliare solamente pezzi residuali della nostra azione parlamentare ad un settore che è fondamentale per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Credo di poterlo e doverlo reclamare a nome del mio Gruppo, e, se me lo consentono, anche a nome di tutti i valorosi senatori "agricoli" che lavorano con me ogni giorno in Commissione agricoltura.

avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Informo l'Assemblea che il Segretario generale del Senato mi avverte che il Presidente è in contatto con la Farnesina, per vedere come

Colleghi, con il voto delle mozioni sono esauriti gli argomenti della settimana, salvo il sindacato ispettivo che resta confermato per domani pomeriggio alle ore 16. Pertanto, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Quel che occorre fare - e il senatore D'Alia lo ha già detto, non sapendo che in Italia non c'è un ambasciatore iraniano, ma un incaricato d'affari - è comunque convocarlo, senza dargli la dignità di riceverlo come membro di Governo,

l'inaccettabilità della reazione violenta nei confronti di chi dissente verso questo regime fascista.